L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. Avverte

lettera del Presidente della Repubblica riguardante il noto decreto milleproroghe, ne ha subito informato l'Assemblea, dandone lettura.

sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione: n. 1, dei senatori Gasparri e Bricolo; n. 2, della senatrice Finocchiaro e di altri n. 3, dei senatori D'Ubaldo ed altri, n. 4, dei senatori Stradiotto ed altri, n. 5, dei senatori Morando ed altri, n. 6, dei senatori Barbolini ed altri,

al grado di autonomia che s'introduce con questo decreto legislativo, ripeto quanto detto nell'intervento di ieri: questo è il massimo livello di autonomia che si può raggiungere senza la tassazione della prima casa,

Signor Presidente, cinque minuti non saranno sufficienti per mettere in fila tutte le ragioni per le quali siamo contrari allo schema di decreto Tuttavia, proverò ad utilizzare il tempo a disposizione per argomentare almeno dieci no a questo provvedimento. Primo "no": non si prevede affatto alcuna responsabilità fiscale degli amministratori nei confronti degli amministrati. Altro che raddrizzare alberi storti. La quota maggiore delle risorse per i Comuni arriverà da compartecipazioni e dal fondo perequativo (cioè da trasferimenti); la stessa IMU, cioè la principale tassa comunale, non riguarderà i residenti-elettori ma solo i non residenti e le imprese. La retorica federalista del principio di responsabilità come strada privilegiata per l'efficienza in questo testo è praticamente assente. Secondo "no": in questa riforma non esiste alcuna semplificazione dell'amministrazione locale (aggregazione dei Comuni, riduzione dei livelli di governo, specificazione o specializzazione delle funzioni): semplicemente, verranno ridotti i servizi, senza migliorare né organizzazione né costi. Terzo "no": il sistema proposto non assicura la copertura finanziaria del fabbisogno dei Comuni. L'addizionale IRPEF e le altre nuove tasse (di soggiorno, di scopo) non andranno a finanziare ulteriori servizi aggiuntivi, ma serviranno solo a coprire il fabbisogno ordinario. Quarto "no": questo federalismo municipale aumenterà la pressione fiscale. Si sta tentando di realizzare una riforma non riducendo la spesa dello Stato e trasferendo, di rimando, quote di potere fiscale a Regioni e Comuni, ma, semplicemente, lasciando ai Comuni licenza di imporre nuove tasse per compensare i pesanti tagli già effettuati da questo Governo al sistema delle autonomie locali. Quinto "no": questo federalismo colpisce le imprese con la stangata dell'IMU. Rispetto all'attuale ICI, l'imposta applicata agli immobili destinati alla produzione sarà quanto meno raddoppiata. Sesto "no": questo meccanismo della cedolare secca non combatte affatto l'evasione, perché non innesta alcun contrasto di interesse tra proprietario e locatario. Settimo "no": è profondamente iniquo proporre una riduzione del 20 per cento per i proprietari senza prevedere significative agevolazioni fiscali per gli inquilini. Altro che sostegno alle famiglie più bisognose! Ottavo "no": il complesso della redistribuzione fiscale contenuta in questo decreto va in una direzione precisa: quella di più tasse per famiglie e imprese, meno tasse sulle rendite. il meccanismo di riequilibrio o di perequazione previsto presenta una preoccupante ed incerta definizione della copertura finanziaria. Resta, dunque, particolarmente oscuro come si realizzerà la perequazione. Decimo "no": il testo in esame è evidentemente esposto ad un giudizio di incostituzionalità e rischia di generare correlate incertezze e precarietà nell'intero sistema della finanza locale. Non mi voglio abbandonare a tecnicismi; tuttavia ricordo che la procedura prevista per l'emanazione dei decreti delegati attuativi del federalismo fiscale costituisce criterio direttivo della delega stessa. Il rispetto di quella procedura è quindi condizione della legittimità costituzionale dei decreti. In questo caso, invece, siamo davanti ad una palese violazione della legge, che ignora persino il richiamo del Presidente della Repubblica in merito alla necessità che questa riforma sia attuata con il massimo della condivisione e del coinvolgimento del Parlamento

Continuo a pensare che sia viziato nella sua genesi. Nonostante le parole del Ministro, e forse anche oltre la sua stessa volontà, questo federalismo nasce dal tentativo di separare il Paese. Credo che tutto ciò sia profondamente sbagliato. L'Italia unita riesce a stento a mantenere un ruolo nel mondo globalizzato. S'illude chi pensa che il Nord d'Italia da solo sia più forte, più competitivo, più sicuro, più stabile. Purtroppo, questo tipo di federalismo, di cui il provvedimento in esame è un tassello importante, è diventato sempre più una bandiera politica. Per tutte queste ragioni, il voto di Alleanza per l'Italia sulle diverse risoluzioni presentate sarà consequenziale agli argomenti appena esposti.

Presidente, signor Ministro per la semplificazione Italia dei Valori ha sempre creduto, e crede ancora, in un'articolazione diversa delle autonomie,

vale a dire di un decentramento che lascia cogliere negli amministratori, per un verso, e negli amministrati, dall'altro, l'essenza vera di un'amministrazione pubblica vicina ai cittadini. È peraltro vero che ci troviamo a a discutere in un'Aula del Parlamento, e dobbiamo rendere grazie al Presidente della Repubblica per aver evitato un colpo di mano del Governo, che aveva approvato un decreto legislativo senza averne i poteri. Siamo tornati quindi a discutere, ad approfondire e a ragionare sugli errori che - a nostro avviso - sono

Innanzitutto, è la negazione della maggiore responsabilizzazione economico-gestionale degli amministratori locali, perché l'autonomia impositiva riservata ai Comuni per tassare le seconde case dei non residenti,

Inoltre, continuiamo a discutere di cosiddetto federalismo fiscale, ma ancora - lo sappiamo bene tutti - non abbiamo la definizione dei fabbisogni standard; ci stiamo cioè arrampicando sugli specchi, perché evidentemente bisogna pagare pegno ad una forza politica che ha fatto del federalismo - non importa se poi tutto il resto dell'azione di governo se ne sta andando a pallino - una bandiera da vendere, magari contro Roma ladrona (anche se il Pio Albergo Trivulzio si trova a Milano, e qualche esponente della Lega è coinvolto anche a Roma

sul testo, cercando di migliorarlo. Vi è poi, a nostro avviso, la grande questione dei numeri, l'impatto finanziario della riforma sui conti dello Stato. Noi riteniamo che non solo non risparmieremo, ma, come diceva ieri il il procuratore generale della Corte dei conti, è verosimile che il sistema corruttivo e, più in generale, il sistema dell'aumento della spesa pubblica possa trovare la sua esaltazione proprio in un federalismo che parta senza la definizione dei costi, senza la definizione dei numeri, come noi abbiamo sottolineato. Riteniamo inoltre che siano state introdotte delle nuove imposte, in questo violando la legge n.

che avrà un impatto depressivo. Ben altro bisognava fare, a cominciare da una riduzione dell'IVA sugli alberghi per riportarla ad una tassazione del 4 per cento, come avviene in altri Paesi dell'Unione europea. Ecco perché noi riteniamo che si

al termine dell'attuazione di tutti i decreti legislativi, la pressione fiscale rimarrà invariata: quindi, nell'anno di mai, nel mese di poi, nel giorno sconosciuto, noi non conosceremo i

un minimo comune denominatore per unire il Paese, non per dividerlo. Noi riteniamo invece che - come d'altra parte, in mancanza di numeri certi, le proiezioni che abbiamo letto

da mettere davvero in condizioni, se non di dissesto, certamente di grave difficoltà il mantenimento dei servizi essenziali. che la cedolare secca che viene introdotta sugli affitti sia fortemente viziata di incostituzionalità, considerando che l'articolo 53 della Costituzione parla di una imposizione progressiva. Noi cosa facciamo invece? La scorporiamo dall'IRPEF, la tassiamo in maniera diversa e, quindi, in maniera proporzionale e non progressiva, favorendo i redditi alti e deprimendo, o quanto meno non avvantaggiando, i redditi più bassi. più bassi. Eravamo e siamo convinti che vi fosse la possibilità di migliorare il decreto, e abbiamo provato a farlo, perché come Italia dei Valori riteniamo che i Comuni debbano avere la possibilità di essere indipendenti e di autodeterminarsi,

Invece, ci troviamo di fronte ad affermazioni di principio. I Comuni, che in un primo momento erano lieti di poter chiudere i bilanci, si rendono conto che dovranno aumentare l'imposizione per mantenere i servizi. Ecco perché abbiamo presentato un

il decreto aumenterà la sperequazione sul territorio, la tassazione dei cittadini e non contribuirà ad una articolazione del territorio che sia davvero al servizio della gente.

non per volontà del Governo e della maggioranza, né per un capriccio dell'opposizione, ma per rispetto di principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, che l'Unione di Centro non ha votato ma che intende rispettare, cioè quella che ha delegato il Governo a lavorare, insieme alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, alla redazione dei decreti attuativi, o meglio dei decreti legislativi, in esercizio della delega conferita dal Parlamento.

Per quale ragione? Per la presunzione di ritenere che anche la legge che la maggioranza ha voluto dovesse essere interpretata in maniera muscolare, e non ancorata ad una procedura che non è solo formale, ma è anche sostanziale. Tale procedura, infatti, di soggetti che compongono la Repubblica, come dice la Costituzione, nella fase di attuazione del federalismo fiscale, e nella Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo reale non vedo un organo tecnico, la camera di compensazione dal punto di vista politico di tutte le questioni che attengono ad una riforma che, per bocca del Governo, dovrebbe essere epocale. Questo è quindi il contesto non dimentichiamolo - nell'ambito del quale stiamo esaminando le comunicazioni del Governo su questo schema di decreto. Il contesto su cui ci muoviamo prende le mosse dal presupposto che la Commissione bicamerale - come incontrovertibilmente definito dal suo regolamento e dalla legge istitutiva - ha respinto la proposta della maggioranza e del Governo. Tutto ciò, signor Presidente, ha una sua incidenza, e lo vorrei dire con assoluta chiarezza. Infatti, con questo decreto si stanno riscrivendo

del procedimento relativo all'adozione di questo schema di decreto potrebbe portare a ricorsi alla Corte costituzionale, alla caducazione del decreto stesso e allo scasso finale dei bilanci dei Comuni del nostro Paese. Di questo bisogna tener conto. E di questo io credo che tutti noi dobbiamo farci carico perché proceduralmente, così come noi abbiamo avuto modo di dire anche in Commissione bicamerale, la via maestra sarebbe stata quella di riattivare il procedimento. Non si può pensare che la Commissione bicamerale sia un orpello che conviene quando è funzionale alle passeggiate mediatiche di qualcuno e, viceversa, quando nel merito pone una serie di questioni, e lo fa con assoluto senso di responsabilità e senza alcuna strumentalità, tutto questo non va bene. Non va bene, non conviene, e quindi è fuori da ogni discussione. Parlo anche senza il Ministro. Non mi offendo. Non è un problema, signor Presidente.

è fondamentale, anche per comprendere come potranno il Governo e questa maggioranza affrontare prove particolarmente complesse che riguardano, dalla nostra prospettiva e dal nostro punto di vista, almeno il 70 per cento della normativa relativa all'attuazione della legge n. 42 del 2009. Vorrei fare due conti per comprendere come la nostra posizione non sia assolutamente strumentale. È vero infatti che abbiamo votato contro la legge n. 42, e lo abbiamo fatto in maniera chiara, sollevando una serie di questioni, di metodo e di merito, soprattutto, che oggi vengono a galla. Emergono nella loro drammaticità, a tal punto che, a maggio, scadranno i 24 mesi per l'esercizio del potere normativo da parte del Governo, e siamo ancora al 30, forse 40 per cento del procedimento di attuazione del federalismo fiscale. Abbiamo da fare altri quattro-cinque decreti legislativi, e tutto questo dovrebbe essere fatto in due mesi, quando non si è fatto in due anni. Ma non è un colpevole ritardo del Governo, non ne faccio carico al Governo: è la condizione economica del nostro Paese. È il sistema istituzionale del nostro Paese che rende oggettivamente complicato poter riscrivere una legge di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, senza incorrere in errori, in contraddizioni e, come avvenuto e avviene nel caso di questo decreto, in atti che sono anche più gravi dal punto di vista della sottrazione dell'autonomia ai Comuni di quanto non sia il sistema legislativo vigente. Questo è il tema di fondo. Allora, la prima questione che abbiamo posto e poniamo con la nostra proposta di risoluzione è questa: come si fa a costruire, ancorché in maniera confusa, con sistemi che tentano di tenere insieme diverse posizioni di di natura ideologica dal punto di vista fiscale, un sistema di autonomia fiscale ed impositiva dei Comuni nuovo quando, per espresso impegno della maggioranza e del Governo, preliminarmente doveva essere esaminata ed approvata la Carta delle autonomie, che riscrive le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Regioni e, in particolar modo, di Comuni, Province ed enti locali? locali? Questo è il punto di fondo. Poiché la Costituzione prevede il principio dell'integrale finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, è altrettanto evidente che l'integralità del finanziamento parte dal presupposto che il legislatore fissi con chiarezza quali sono le competenze dei Comuni, e su quelle, e sulla specificità di quelle funzioni e di quelle competenze, ancora il sistema autonomo dal punto di vista impositivo o fiscale. Tutto questo non c'è, perché la Carta delle autonomie dorme in Parlamento - credo qui in Senato questa è una condizione che rischia di far crollare il sistema che si vuole mettere in piedi. È evidente infatti che quando il sistema fiscale poggia su una definizione provvisoria e forfettaria delle funzioni fondamentali dei Comuni, si dà per presupposto o che non si voglia fare la riforma del sistema delle autonomie locali o che comunque esso dovrà essere cambiato quando cambierà il sistema di competenze e di funzioni delle autonomie locali. La seconda questione, molto chiara,

e riguarda la circostanza che non si può immaginare di costruire un sistema che nella sua fase transitoria attribuisce al centro la maggior parte delle risorse, deresponsabilizzando i Comuni, per consentire una perequazione i cui criteri non sono peraltro noti e non si capisce quali siano, a tal punto che il Governo chiede di espungere dalla nostra proposta risoluzione proprio la parte che lo vincola a definire questi criteri. allora che parte per essere autonomo, decentrato e più libero dal punto di vista degli enti locali, diventa ancor più centralista centralista in ragione del fatto che per poter far quadrare i conti degli enti locali nella fase transitoria, fino a quando non si arriva a regime, bisogna intervenire con questo fondo perequativo transitorio, le cui regole sono note forse a qualcuno, ma certamente non al Parlamento.

le piccole e medie imprese, che sono l'oggetto del desiderio di questa riforma fiscale, vengano o debbano essere trattati dai sindaci come degli extracomunitari.

introiti sul piano della lotta all'evasione, perché ognuno dichiara o non dichiara se si tratta di prima o seconda casa, e così via: sono tutte cose bellissime, principi condivisibilissimi, ma noi in questa sede dobbiamo fare conti, calcoli e numeri, e non possiamo limitarci a dire che faremo, diremo e colpiremo. inoltre sull'imposta di scopo, che è una patrimoniale, perché colpisce ovviamente il patrimonio di tutti per realizzare determinate opere pubbliche, sulla tassa di soggiorno, che riguarda i non residenti, e sulla circostanza che in questo contesto vengano colpite le attività commerciali ed imprenditoriali in misura superiore di quanto non avvenisse prima con la cosiddetta ICI. Tale sistema porta alla logica conclusione che, se autorizziamo anche i sindaci a rilasciare il permesso di soggiorno per i non residenti, probabilmente rendiamo coerente il sistema normativo di cui ci stiamo occupando. Queste sono alcune delle ragioni delle ragioni che ci portano a confermare il nostro no di merito su questa vicenda, perché, così come noi abbiamo detto in quest'Aula, in sede di dichiarazione di voto sul federalismo fiscale, l'unica cosa certa di questa riforma è che i sindaci per far quadrare i bilanci dopo il decreto Tremonti dovranno utilizzare l'addizionale IRPEF, il sistema delle compartecipazioni e ampliare la pressione fiscale, cioè più tasse per tutti. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giacomo Matteotti» di Maerne, in provincia di Venezia. Rivolgiamo loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

La prima era la compartecipazione all'IRPEF; la seconda, l'IMU sulla seconda casa e le attività produttive (in sostanza, un nuovo nome alla vecchia ICI); la terza, una forma di cedolare secca, priva di deduzioni per gli inquilini e, quindi, priva di contrasto di interessi. Ad esse si aggiungevano la tassa di soggiorno e le imposte di scopo.

quantitative dimostravano che, con una simile impalcatura, aumentava il centralismo statalista delle risorse; aumentava il peso del fondo di perequazione e quindi, di fatto, dei trasferimenti; veniva meno il principio del cittadino che paga le tasse e controlla la spesa, come ha appena detto il collega D'Alia (infatti, se a pagare le tasse ai Comuni sono prevalentemente i non residenti, è evidente che quel principio viene meno). Il combinato disposto di tale impalcatura non può che portare più tasse per tutti, per la semplice e banale ragione che, se lo Stato non le riduce e i Comuni le possono aumentare, l'aritmetica indica che si determinerà una maggiore tassazione a carico dei cittadini: che è l'obiettivo perverso del federalismo, perché chi è federalista convinto sa che lo strumento federale, che responsabilizza tutti i livelli di governo, ha come scopo primario quello di controllare la spesa pubblica, di contenerla, ridurla e migliorarla nella qualità dei servizi.

Debbo dire che la conclusione che abbiamo ottenuto è modesta, da questo punto di vista, perché la maggioranza e il Governo si sono convinti che poggiare la compartecipazione sull'IRPEF, che è un'imposta molto più sperequata sul territorio rispetto, ad esempio, all'IVA, poteva essere l'unico aspetto accolto è stato quello di modificare il testo passando dalla compartecipazione IRPEF alla compartecipazione IVA; per gli altri punti, invece, non c'è stata alcuna possibilità di procedere a ulteriori aggiustamenti. in tutti i Paesi federali del mondo la finanza locale dei Comuni poggia su due cespiti; autonomi e specifici: i consumi da una parte (negli Stati Uniti d'America si chiama *sales tax*, mentre in Europa e in Italia si chiama IVA) e gli immobili dall'altra. È evidente che tale sperequazione, anche in termini di controllo del cittadino che paga le tasse e ottiene i servizi,

che è stato realizzato in precedenza quando si azzerò l'ICI sulla prima casa da parte del Governo Prodi e poi del Governo attuale. Con quell'obbrobrio, in realtà, si è tolto uno dei pilastri del federalismo comunale.

che il cittadino paga l'IMU sulla prima casa al Comune detraendola completamente e istantaneamente dall'IRPEF. Sarebbe un'operazione

permetterebbe di riequilibrare enormemente il gettito dei Comuni, ridurrebbe il ruolo del fondo di perequazione e quindi riequilibrerebbe in termini corretti il federalismo fiscale municipale. È evidente, infine, signor Presidente, che

che è quella di mirare all'emersione degli affitti in nero. È inaccettabile, lo ripeto in quest'Aula, che ci sia un bollino della Ragioneria generale dello Stato che certifica 3 miliardi di recupero di affitti in nero

una certificazione della Ragioneria generale dello Stato per ben 3 miliardi, che improvvisamente apparirebbero in questo anno 2011 come frutto dell'emersione degli affitti in nero

ha annunciato, intenderà proseguire su questa strada, impegnandosi a correggere le distorsioni che l'impalcatura che abbiamo di

se non si fanno questi aggiustamenti, il ruolo del fondo di perequazione aumenta, ma se non funziona il fondo di perequazione, il Paese si spacca.

confermare alcuni indirizzi di principio di questo provvedimento, per esempio quello sul non incremento della pressione fiscale, che costituisce una vero *leit motiv*, una sorta di *slogan* che ispira tutta l'azione politica non tanto del Governo, quanto della forza politica che ne ha acquisito la *leadership* sostanziale, cioè la Lega. c'è tutta la forza politica, la capacità di imprimere a questo Governo una *ratio*, poiché altre non ne ravviso: quella di fare il federalismo, che è la ragione vera di sopravvivenza di un Esecutivo segnato da condizioni di debolezza strutturale assolutamente evidenti. La Lega è garante del Governo e questo provvedimento è la sostanza stessa della sua funzione politica. per queste ragioni il provvedimento supera il merito e assume un valore simbolico, e la procedura che è stata definita per l'approvazione di questo testo è il segno più evidente di questa condizione particolare.

Il decreto milleproroghe segue la vicenda del decreto sul federalismo municipale. Non è più un caso se il Presidente della Repubblica deve intervenire costantemente per richiamare l'Esecutivo a un rapporto diverso con il Parlamento.

ha enunciato in modo assolutamente preciso. Per questa ragione ci attestiamo su una linea critica verso il provvedimento

senza definire prima i fabbisogni standard. Ho ascoltato poc'anzi - ed è stata un'opportunità molto positiva - l'intervento del collega Baldassarri, che ha rivendicato questa correzione di rotta dalla compartecipazione IRPEF alla compartecipazione IVA. Anche in

potenzialmente divaricante rispetto ai diversi territori. Anche l'opportunità prevista all'interno della cedolare sugli affitti è stata gestita in termini non condivisibili. La scelta della proporzionalità, rispetto alla progressività dell'imposta, ovviamente non è equa e si caratterizza per un favore naturale che questa coalizione rivolge ai ceti più abbienti.

- sostiene la necessità di alcuni emendamenti indispensabili per non violare le prerogative statutarie. Ho ascoltato ieri il ministro Calderoli che, con un passaggio cortese e rassicurante, ha detto

È un percorso ineluttabile, che vuole tutto il Paese, che chiedono tutti i sindaci e gli amministratori locali per risolvere gli antichi guai del rapporto tra Stato e autonomie, per dare attuazione alla Costituzione e mettere sullo stesso piano i vari livelli della pubblica amministrazione, per suggellare i principi di autonomia e responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Tutto il Paese potrà trarre beneficio da questi nuovi strumenti, tanto chi è già pronto quanto, e forse di più, chi deve recuperare il terreno perduto nelle sabbie dell'assistenzialismo e dell'inefficienza. Per questo non credo ai mille distinguo di chi dai banchi dell'opposizione dileggia questo processo. Non siamo nuovi a questo messaggio. Lo abbiamo già visto nel 2005-2006, in occasione di un'importante riforma costituzionale che avrebbe cambiato il bicameralismo perfetto, ridotto il numero dei parlamentari, riordinato in maniera efficiente le competenze delle Regioni. per voler dire che si deve fare di più e di meglio, qualcuno come allora esprime contrarietà a questi provvedimenti.

come stampella del riformismo, ma a condizione di far cadere il Governo in carica. Quale obiettività nel merito possono avere queste proposte, di fronte alle richieste pressanti delle autonomie? Questa riforma non è né di destra, né di sinistra, e non deve dipendere da questo o da quel Governo. Ma avete ascoltato, letto, colto le richieste dei Comuni, delle Province e delle Regioni, i pareri e i contributi che hanno formulato ai vari testi che si sono succeduti in Commissione? Non solo, ma mi sembra che questa *verve* propositiva non si sia sempre concretamente manifestata nei lavori della Commissione. Caso mai, in questi ultimi mesi, abbiamo dovuto ascoltare, a proposito di pressione fiscale, le più disparate proposte, da parte di alcuni importanti esponenti della sinistra di governo, a a proposito di soluzioni fiscali e interventi risolutori del gravame del debito pubblico. Ricordate l'onorevole Amato, che ha proposto a un terzo degli italiani di pagare 30.000 euro a testa

Dimenticate queste proposte? Questo federalismo garantisce invece, a parità di pressione fiscale, una maggiore autonomia agli enti locali. L'insieme delle compartecipazioni consente un legame diretto tra le imposte relative agli immobili e i Comuni. E la riformulazione dell'imposta municipale propria, così come dimostrato dalle proiezioni,

Allora, signori, il lupo perde il pelo, ma non il vizio: soprattutto quello di mistificare la realtà. Vi chiedo un ulteriore sforzo di memoria, ma questo è molto più recente, e quindi non possiamo dire di esserci già dimenticati. Ho qui un piccolo studio

L'emendamento 23 (a firma Boccia) portava la cedolare secca al 23 e al 18 per cento: costava alla collettività 578 milioni di euro in più. l'incremento della componente aggiuntiva IMU da 20 a 150 euro: costava al contribuente da 1,2 fino a 8,9 miliardi di euro. L'emendamento 50 (Vitali)

la proposta di federalismo municipale che sarebbe stata accolta e voluta dal centrosinistra e dal Partito Democratico? Ho tralasciato poi la famosa proposta della *service tax*, di cui tanto avete parlato, che reintroduceva surrettiziamente l'ICI sulla prima casa,

magari dopo anni e anni di onerosi finanziamenti bancari. È questa la politica di contenimento della pressione fiscale che avreste attuato con il vostro federalismo municipale?

fate queste proposte e poi dite che siamo noi ad incrementare la pressione fiscale. E invece, grazie a questo federalismo municipale, la pressione fiscale rimarrà invariata e i Comuni avranno risorse proprie. Sulla base di queste semplici ed evidenti motivazioni,

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo sperato fino a questa mattina che il suo parere cambiasse rispetto alla possibilità di modificare lo schema convinti che i Governi cambiano, passano, ma le riforme restano. In questo senso sono certo, siamo certi, che se questo Parlamento fosse stato eletto

si basa su alcuni principi fondamentali: autonomia finanziaria di entrata e di spesa, risorse autonome e tributi ed entrate proprie. Il federalismo che voi proponete non ha nulla di questo: si tratta solo di finanza derivata, che arriva dall'alto ed è decisa dall'alto.

perché non ci sono di fatto i tributi propri: l'IMU è un imposta che pagheranno solo quelli che in un dato Comune non votano, perché hanno la seconda casa o hanno la proprietà dell'attività produttiva, ma non è detto che nel Comune stesso abbiano la residenza e quindi

e le spese che in quel territorio vengono sostenute, perché questo incentiva il senso civico e la lotta all'evasione. La lotta all'evasione non si fa solo ed esclusivamente con la Guardia di finanza ma soprattutto e innanzitutto investendo sul senso civico.

Ma chi è che paga l'IRPEF in Italia? L'IRPEF è quell'imposta che pesa per l'85 per cento sulle spalle di lavoratori dipendenti e pensionati:

anche sulla leva dell'ICI; quindi, un sindaco, un consiglio comunale avevano la possibilità di modulare quel prelievo. Oggi, i tagli determinati dalle varie finanziarie che avete il Patto di stabilità perverso che avete applicato e che strozza i Comuni, sommati ad una situazione economica più difficile di qualche anno fa impongono di fatto che l'addizionale IRPEF diventi l'unica valvola di sfogo.

PD)*. Questa non è autonomia! Questo non è federalismo! Il « pago, vedo, voto» non esiste, come ho avuto modo di sottolineare in precedenza: è tutta finanza derivata. un sistema assolutamente confuso e complicato, mentre la semplificazione è la base essenziale per il funzionamento di un sistema fiscale. Il cittadino deve capire dove vanno a finire i suoi soldi; invece i soldi continueranno

un'occasione e state facendo una cattiva riforma. Siete dei bravissimi venditori di fumo: su questo non vi batte nessuno! Il tempo, però, è galantuomo e la verità salterà fuori. Tra qualche mese, quando il fumo sarà diradato, emergerà più chiaramente la realtà. Non credo che potrete più scrivere sui manifesti elettorali: «padroni a casa nostra»;

e ci dispiace veramente che non abbiate accolto le nostre proposte, volte alla riduzione delle tasse per gli onesti. Noi, caro senatore Franco, proponevamo l'abolizione dell'addizionale IRPEF, perché quella è una cosa seria: abbassare veramente la pressione fiscale, un abbassamento delle imposte per le imprese, un abbattimento degli sprechi e soprattutto una grande lotta all'evasione fiscale. Concludo, signor con un appello al ministro Calderoli. Vede, ministro Calderoli, l'anno scorso, a Pontida, ha iniziato il suo discorso facendo riferimento all'Italia e dicendo che la nave prima di affondare si spezza. Ebbene, non so se quella fosse una preoccupazione o un auspicio. Se era una preoccupazione, questo decreto non risolve quei problemi; se invece era un auspicio, comprendo perché l'avete fatto così, e per questo noi voteremo assolutamente contro.

*(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, (almeno per ciò che concerne i Comuni) l'anello di un processo di profonda trasformazione in senso federale della pubblica amministrazione e delle autonomie locali, che a partire dalla legge delega n. 42, attraverso i decreti sul federalismo demaniale e sui costi e fabbisogni standard, si è dipanato in questi due anni di lavoro. Un percorso normativo che colma un vuoto legislativo ormai ultradecennale, più volte deprecato dalla Corte costituzionale: un vuoto che ha, fino ad oggi, impedito il pieno dispiegamento degli effetti delle riforme costituzionali del 1999 L'impellere della crisi economica mondiale, la crisi cronica della pubblica amministrazione italiana, impastoiata fra inefficienze, sprechi e il perdurare di fenomeni di corruzione, la conseguente crisi di consenso politico sono tutti fenomeni che hanno impresso una sensibile accelerazione al federalismo. È oggi più che mai evidente la necessità di riavvicinare la pubblica amministrazione al cittadino, di riunire i due capi del filo che corre dal prelievo tributario alla spesa pubblica, di perseguire il principio della responsabilità diretta nella gestione delle risorse. La stessa ANCI ha riconosciuto che il federalismo, declinato correttamente e autenticamente, (ossia garanzie di copertura finanziaria, con entrate autonome, del fabbisogno delle funzioni pubbliche assegnate sulla base di standard e integrate con le risorse perequative, accompagnato da piena e responsabile autonomia complessiva di spesa che consenta anche di sostenere la crescita dei territori) rappresenta la soluzione possibile e forse unica per risolvere i problemi del comparto delle autonomie locali. Il processo federale ha indubbiamente il pregio di introdurre elementi aziendalistici nella gestione pubblica, attraverso meccanismi di tariffazione delle prestazioni erogate, non dissimilmente da quanto già accaduto nel campo della sanità. La riforma ha il pregio di affrontare in modo frontale il problema della ripartizione ottimale delle risorse, ma anche il tema delle inefficienze e degli sprechi della pubblica amministrazione.

Si apre oggi la strada ad un processo di aziendalizzazione della cosa pubblica che ha mosso i suoi primi passi negli anni '90, con esiti non uniformi sul comparto pubblico. Il comparto degli enti locali, nonostante la pur forte accelerazione impressa al decreto legislativo n. 77 del 1995, ha segnato fino ad oggi il passo. La riforma poggia, senatore Garraffa, il percorso di ricerca dell'efficienza...

*(PdL)*. La riforma poggia il percorso di ricerca dell'efficienza sul cardine dei livelli essenziali delle prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale in analogia ai livelli essenziali di assistenza (LEA) che sono il cardine del Sistema sanitario nazionale ed il fulcro dei processi di federalismo sanitario. L'altro cardine della messa in efficienza del sistema è la rilevazione dei costi standard, un nuovo modello di finanziamento basato sui costi di produzione delle singole prestazioni. Di più, il legislatore introduce il concetto del «fabbisogno standard» quale «costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficacia e l'efficienza costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica». Una rivoluzione copernicana del sistema in grado di assicurare, a regime, il definitivo abbandono del sistema della spesa storica, che fino ad oggi ha perpetuato inefficienze e sprechi, senza mai introdurre, se non residuali, elementi di premialità. È l'avvio di un sistema di analisi dei bisogni che imporrà ai Comuni uno sforzo di mappatura delle necessità espresse dalla collettività: un percorso che porterà a standardizzare i fabbisogni ed i costi dei servizi da erogare. D'altra parte, il sistema di perequazione introdotto dalla riforma assicura il rispetto del principio costituzionale di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione, declinando l'articolo 119 che fa esplicito riferimento ai «territori con minore capacità fiscale per abitante». Quali sono i punti di forza di questo progetto? Si introducono principi di responsabilizzazione degli amministratori; e Dio sa quanto c'è bisogno di responsabilizzare gli amministratori, che negli anni scorsi hanno utilizzato le risorse pubbliche soltanto per eventi di natura ludica e non per pensare agli effetti sul territorio! È avvenuto anche nella nostra Sicilia, senatore Garraffa. Si tende all'aumento dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, vera chiave di volta del federalismo. E in questa riforma vi è l'autonomia impositiva da parte dei Comuni, come è stato abbondantemente dimostrato dal Ministro e dagli interventi dei senatori della maggioranza. La semplificazione normativa, attraverso l'accorpamento di oltre 45 tributi stratificatisi ed a vario titolo gravanti sulle medesime fattispecie implementa il divieto di doppia imposizione sulla medesima fattispecie imponibile, declamato dalla legge delega, al fine di evitare che moltiplicando i soggetti impositori aumenti anche il peso fiscale sul medesimo bene. In particolare, le modifiche apportale all'originario schema di decreto, introducono diverse innovazioni di pregio. Per quanto riguarda le compartecipazioni, oltre a quelle già individuate, di cui viene quantificata la quota di spettanza dei Comuni: il 30 per cento dei proventi dei tributi immobiliari e quella relativa alla cedolare secca, ora fissata al 21,7 per cento e per il 2012 al 21,6 per cento, viene adottata anche la compartecipazione all'IVA prodotta nel territorio. La novità è introdotta sulla base dell'esperienza empirica e dei dati analitici i quali confermano che la distribuzione dell'imposta sui consumi è meno sperequata fra Nord e Sud di quanto non lo sia quella quella sui redditi. In questo modo si tende a garantire una forma di perequazione alle aree più svantaggiate del Paese. Ancora, viene data centralità al fondo sperimentale di riequilibrio, che per tre anni garantirà gli equilibri finanziari dei Comuni. Si introduce il criterio demografico per una quota parte pari al 30 per cento della dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio. Si introduce una norma in favore degli inquilini attraverso il blocco per l'intera durata dell'affitto dell'adeguamento automatico del canone, anche quello relativo all'aggiornamento ISTAT, in ipotesi di esercizio della facoltà di applicazione della cedolare secca sugli affitti, che dovrà essere comunicata con lettera raccomandata agli inquilini stessi. Si introduce la facoltà per i Comuni di istituire l'imposta di soggiorno, variabile fino ad un massimo di 5 euro per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva e di riutilizzare le risorse per interventi in materia turistica, nonché di potenziamento del trasporto pubblico locale: norma che se sapientemente e prudentemente usata, non essendo per l'esiguità degli importi tale da turbare gli equilibri dei flussi turistici, può contribuire ad indirizzare risorse nuove verso lo sviluppo turistico dei territori. Di capitale rilevanza è la questione relativa alla lotta all'evasione fiscale, attraverso il potenziamento del ruolo dei Comuni, poiché il decreto, oltre a mettere a disposizione dei Comuni l'anagrafe tributaria, stabilisce che il 50 per cento (prima era il 33 dei tributi recuperati verrà devoluto ai Comuni e, allo stesso tempo, che le sanzioni per chi non abbia dichiarato le abitazioni fantasma verranno quadruplicate. Il 75 per cento delle entrate

conseguente ad un miglioramento dell'efficienza per effetto dell'applicazione dei fabbisogni standard e di una migliore riallocazione delle funzioni tra i livelli di governo, e che è esplicitamente previsto operi in regime di invarianza della pressione fiscale. Alla luce di tutte le superiori considerazioni che trovano puntuale riscontro nel decreto legislativo - che è stato anche apprezzato da tutti i sindaci dei Comuni riuniti nell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia lo stesso chiaramente rappresenta un primo e importante passo in un percorso virtuoso, se pur difficile, di rifondazione del sistema delle autonomie locali. Ecco perché il Popolo della Libertà, tramite me, annuncia il voto favorevole alla proposta di risoluzione

Signor Presidente, capisco l'apertura del Governo e della maggioranza, però però noi chiediamo anche un impegno sul periodo transitorio, che non riguarderà chissà quale esercizio ma l'esercizio 2011, 2011, un esercizio già avviato. La perequazione così come consegnata da questo provvedimento, entra già in crisi adesso. Il risultato - noi temiamo

ho già detto prima in dichiarazione di voto rispetto all'intero provvedimento - la necessità di dare più autonomia e responsabilità ai Comuni e agli amministratori locali,

e questo soprattutto per l'esercizio dell'attività di impresa, di professione e di lavoro autonomo in generale. Chiediamo alla maggioranza ed al Governo un ripensamento su questo punto e chiediamo di rendere obbligatorio il dimezzamento dell'IMU

continuano a considerare differente dai numeri, che in molti caso mancano, e da quelli che si stanno facendo strada. Segnalo al Ministro della semplificazione il vero dramma del processo che lui sta portando avanti è quello di un'ulteriore complicazione burocratica ed amministrativa. Questa sarà materia per una battaglia nel Paese: aumentano le tasse, cresce la complicazione burocratica,

Colleghi, stiamo lavorando correttamente e serenamente, anche perché si tratta di un passaggio delicato. Gradirei che si scandissero anche le votazioni e che ognuno possa dire la propria in occasione delle votazioni.

come l'ipotesi di applicazione della cedolare secca abbia assolutamente bisogno, per determinare l'emersione di gettito auspicata, del contrasto d'interessi e quindi di una misura che consenta agli inquilini di dedurre una parte del canone d'affitto.

La cedolare secca, così come è impostata, favorisce i redditi elevati e mortifica e penalizza le fasce più deboli della popolazione. Noi abbiamo bisogno, e in questo senso abbiamo avanzato tale proposta, che si introduca un meccanismo perequativo, avendo anche riguardo al tema della salvaguardia dell'istituto dei canoni concordati per le aree ad elevata densità abitativa, che rischiano di essere di essere messi in un cono d'ombra che accentuerà le difficoltà che poi andranno a scaricarsi sui Comuni. Per tali ragioni e per un'assunzione di responsabilità di fronte al Paese, perché fra qualche tempo vedremo il risultato di questa proposta e di tale misura, chiedo la votazione mediante

contiene esattamente il principio che lo stesso Ministro ha diffusamente illustrato nella sua relazione, cioè che sulla

che sono state puntualmente spiegate. Questa proposta di risoluzione prevede una soluzione molto semplice, che poteva proporre lo stesso Governo (e francamente non riesco a comprendere come non si accolga una misura di questo tipo), inserire nell'emanando decreto legislativo, o in altri provvedimenti correttivi, presìdi chiari per evitare l'aumento della pressione fiscale complessiva. Il Governo dice di no anche a questa proposta? pure, ma non venga a raccontare a noi e, soprattutto, al Paese che non sta operando per l'aumento della pressione fiscale, perché invece sta operando per l'aumento delle tasse per tutti.

nell'apprezzare lo sforzo di grande dinamismo e impegno del ministro Calderoli e la sua straordinaria capacità di far quadrare il cerchio, che in realtà siamo riusciti a varare un'ipotesi di decreto delegato al termine della quale avremo ucciso il sistema delle autonomie, avendo anche il coraggio di chiamarlo federalismo. sostanzialmente, cerca di rimediare e di lanciare un allarme adeguato al sistema delle autonomie.

espresso sulla proposta di risoluzione dei senatori Baldassarri ed altri, preciso che l'orientamento favorevole del Governo è subordinato alla riformulazione della proposta nel senso di espungere le premesse, nonché di modificare i primi quattro punti della parte dispositiva. Il primo e il secondo punto dovrebbero essere unificati, e al contempo occorrerebbe precisare che gli impegni indicati al Governo relativi ad interventi di maggior tutela verso le famiglie locatarie di abitazioni dovranno trovare attuazione nei prossimi schemi di decreto legislativo. Il terzo punto dovrebbe essere riscritto affinché il Governo sia impegnato a prevenire eventuali aggravi fiscali complessivi ricadenti sulle attività imprenditoriali a causa dell'istituzione di un'imposta municipale propria.

al dovuto rispetto delle istituzioni che prendono parte all'*iter* di esame e delle sedi parlamentari e a prevedere nei prossimi schemi di decreto legislativo interventi di maggiore tutela verso le famiglie locatarie di abitazioni, in particolare quelle con più figli; a prevenire eventuali aggravi fiscali complessivi ricadenti sulle attività imprenditoriali a causa dell'istituzione dell'imposta municipale propria; a rendere noti i criteri mediante i quali verrà utilizzato il Fondo sperimentale di equilibrio (che sostituirà i trasferimenti) e come verrà ripartito tra i Comuni; a prevedere meccanismi di "contrasto di interessi" tra locatori e conduttori in modo da rendere più efficace e perseguibile l'obiettivo di impedire l'evasione fiscale nelle locazioni immobiliari».

svolto con il ministro Calderoli e, come avevo già anticipato, intendo chiedere il voto per parti separate per valutare dove c'è la convergenza, possibilmente ampia, su questo dispositivo.

chiederei di mettere ai voti separatamente le tre parti, in modo che l'Assemblea valuti la più ampia convergenza sui punti che riguardano gli impegni di Governo, salvo poi distinguerci sulle valutazioni più politiche relative al testo

vi è una frase che riguarda il fondo di perequazione che non è oggetto di riformulazione, ne chiediamo comunque la votazione. Questo ha detto il presidente Baldassarri. Mi sembra una posizione accettabile perché il testo riformulato dal Governo non riguarda quel punto della perequazione, cioè la seconda parte del punto terzo del dispositivo di risoluzione. Quindi credo che sia assolutamente legittimo chiederne la votazione per parti separate. Però, in presenza di non condivisione unanime, la Presidenza ha il dovere di mettere ai voti la richiesta. Non è la prima volta. Quindi non posso farne a meno. Senatore

Queste vicende sono superate da una dichiarazione del Gruppo dei colleghi del Popolo della Libertà contraria alla riformulazione che il Governo ha proposto all'Assemblea, dice che vogliono che si voti il testo originale della proposta di risoluzione. A questo punto, sarebbe opportuno comprendere quale sia l'opinione del Governo: se intende mantenere la riformulazione o ritirarla. Non può chiedere a noi di di ribadire una posizione che già abbiamo assunto in un dialogo che abbiamo avuto con il Governo. È successiva a questo fatto la dichiarazione dei colleghi del PdL che dicono di essere contrari a che si metta ai voti la riformulazione del Governo.

del parere del Governo, ritirare la premessa, sulla quale vi è parere contrario, accettare la riformulazione della parte

e accetta che si voti sulla riformulazione del dispositivo, credo che facciamo un buon lavoro, perché, in effetti, questo dispositivo contiene valutazioni e conclusioni del tutto apprezzabili. Signor Presidente, le chiedo scusa, ma forse non riesco a capire bene. Abbiamo fatto un lavoro con il Governo, che ha proposto una riformulazione della parte impegnativa che noi condividiamo; a seguito di questo, mi sono permesso di chiedere la votazione per parti separate,

Mi pare che il Popolo della Libertà abbia chiesto di votare non quanto concordato con il Governo, o comunque la parte del dispositivo, ma di tornare a votare l'iniziale stesura della proposta di

che intende dare parere favorevole solamente sulla riformulazione del dispositivo, a prescindere dalla premessa. Se il senatore Baldassarri ritira la premessa, noi non abbiamo alcun problema; se invece non vuole ritirare la premessa, così come il Governo ha espresso la sua contrarietà noi ribadiamo la stessa contrarietà alla votazione per parti separate.

Ad ogni buon conto, mantengo la mia richiesta di votazione per parti separate, perché sul dispositivo c'è consenso, ed è bene che l'Aula si esprima con un ampio consenso, e nella discussione dei testi c'è l'identità politica.

bandiera tricolore, nell'inno nazionale ed in Roma capitale i simboli fondamentali dello Stato repubblicano e del patrimonio dei valori nazionali riconosciuti nel resto della Carta costituzionale,

Non vi è una prassi consolidata di leggere tutte le note che il Presidente della Repubblica inoltra ai Presidenti dei due rami del Parlamento, anche perché nella giornata di ieri questa Presidenza ha tempestivamente inoltrato ai Capigruppo copia della nota affinché ne avessero notizia, loro e, naturalmente, i componenti dei loro Gruppi. Per evitare qualunque possibilità di fraintendimento circa la trasparenza che questa Presidenza intende garantire all'Aula, e quindi per evitare polemiche del tutto infondate, questa Presidenza ritiene di dare lettura della lettera del presidente Napolitano, senza aprire alcun dibattito, perché sulle lettere del Presidente della Repubblica non si apre dibattito. Le lettere del Presidente della Repubblica si ascoltano

ho attentamente esaminato i contenuti delle modifiche e delle aggiunte apportate, nel corso dell'esame al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto‑legge 29 dicembre 2010, n. 225,

ed assegnato alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio il 7 gennaio 2011. L'esame in sede referente, iniziato il successivo 19 gennaio, si è concluso l'11 febbraio, con l'approvazione di 104 emendamenti. Nello stesso giorno è iniziato l'esame in Assemblea, che si è concluso mercoledì 16 febbraio con l'approvazione del maxiemendamento presentato dal Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, che riproduce il testo delle Commissioni con l'aggiunta di numerose altre disposizioni. L'esame in prima lettura ha dunque consumato 50 dei 60 giorni tassativamente previsti dalla Costituzione per la conversione in legge dei decreti‑legge nonostante che l'esame nell'Assemblea del Senato si sia concentrato in pochi giorni. A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni del Senato e dal Governo con il successivo maxiemendamento, al testo originario del decreto-legge, costituito da 4 articoli (di cui il terzo relativo alla copertura finanziaria e il quarto all'entrata in vigore) e 25 commi, sono stati aggiunti altri 5 articoli e 196 commi. Molte di queste disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione. ciò è avvenuto nonostante l'intendimento manifestato dal Governo al Capo dello Stato in sede di illustrazione preventiva del provvedimento d'urgenza, poi confermato con l'approvazione del testo da me successivamente emanato, di limitare a soli tre mesi le proroghe non onerose di termini in scadenza entro il 31 dicembre 2010, rendendo facoltativa la ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 di quei termini e degli altri indicati in apposita tabella attraverso l'eventuale adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; nonché di prevedere pochi e mirati interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. È appena il caso di ricordare che questo modo di procedere, come ho avuto modo in diverse occasioni di far presente fin dall'inizio del settennato ai Presidenti delle Camere e ai Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, si pone in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15, comma 3, della legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, recepiti dalle stesse norme dei regolamenti parlamentari. L'inserimento nei decreti di disposizioni non strettamente attinenti ai loro contenuti, eterogenee e spesso prive dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, elude il vaglio preventivo spettante al Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti-legge.

Tali considerazioni sono state da me ribadite ancora di recente con la lettera in data 22 maggio 2010 inviata in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 in materia di incentivi, recante le norme anti-evasione di contrasto alle c.d. frodi-carosello. Sono consapevole che una eventuale decisione di avvalermi della facoltà di richiedere una nuova deliberazione alle Camere del disegno di legge in esame ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per il momento in cui interviene a seguito della pressoché integrale consumazione da parte del Parlamento dei termini tassativamente previsti dall'articolo 77 della Costituzione, potrebbe comportare la decadenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge da me emanato nonché di quelle successivamente introdotte in sede di conversione: ed è questa la ragione per la quale vi sono solo due precedenti in cui tale facoltà è stata esercitata nei confronti di disegni di legge di conversione di decreti-legge dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996 che ha ritenuto di norma costituzionalmente illegittima la reiterazione dei decreti-legge (entrambi da parte del Presidente Ciampi, che in data 29 marzo 2002 e 3 marzo 2006 chiese una nuova deliberazione alle Camere sulle leggi di conversione dei decreti-legge 25 gennaio 2002, n. 4 e 10 gennaio 2006, n. 2). Devo osservare peraltro che l'ordinamento prevede la possibilità di ovviare a tali inconvenienti, attraverso sia la regolamentazione con legge dei rapporti giuridici sorti sulla base del testo originario del decreto, sia la riproposizione in uno o più provvedimenti legislativi, anche di urgenza, di quelle disposizioni introdotte in sede di conversione che si ritengano conformi ai princìpi costituzionali. allorché, come in questo caso, la decadenza del decreto-legge sia riconducibile al rinvio del disegno di legge di conversione in legge ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, anziché alla mancata conversione da parte delle Camere nei termini stabiliti dall'articolo 77, ritengo possibile anche una almeno parziale reiterazione del testo originario del decreto-legge. Ho ritenuto di dovervi sottoporre queste considerazioni perché a mio avviso non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento da un lato e fra maggioranza ed opposizione dall'altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati. Mi riservo altresì, qualora non sia possibile procedere alla modifica del testo del disegno di legge approvato dal Senato, di suggerire l'opportunità di adottare successivamente possibili norme interpretative e correttive, qualora io ritenga, in ultima istanza, di procedere alla promulgazione della legge. Devo infine avvertire che, a fronte di casi analoghi, non potrò d'ora in avanti rinunciare ad avvalermi della facoltà di rinvio, anche alla luce dei rimedi che l'ordinamento prevede nella eventualità della decadenza di un decreto-legge, come ho sopra ricordato». Mi permetto di aggiungere che la Presidenza del Senato si rende garante dell'applicazione rigorosa dei suggerimenti dati dal Capo dello Stato con questa lettera. *(Applausi).*

Lo scorso anno ci siamo trovati a metà settembre a prendere in considerazione un documento che era stato licenziato in primavera. Oggi siamo al 23 febbraio

Senatore Casson, Signor Presidente, volevo intervenire per segnalare una situazione e per sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni. Voglio parlare della crisi degli stabilimenti produttivi della società Vinyls di Porto Marghera, di Ravenna e di Porto Torres.

che con gli stipendi di febbraio 2011 si rischia di esaurire tutte le ultime disponibilità. Questa situazione di grave crisi era stata segnalata dai senatori del Partito Democratico già all'inizio del 2010. In particolare, con una prima interrogazione

e al Ministro della giustizia, era stato chiesto di sapere quali fossero le previsioni di carattere economico-finanziario, come i Ministri in indirizzo intendessero tutelare i lavoratori inoltre, se essi fossero a conoscenza delle circostanze relative a rischi segnalati di incidente, con particolare riferimento alle segnalazioni di diminuzioni del numero del personale e dei vigili interni allo stabilimento addetti alla prevenzione e alla sicurezza. In quella circostanza, inoltre, erano state chieste notizie al Ministro della giustizia in riferimento ad un procedimento penale per ipotesi di violazione di norme, sia della legge fallimentare,

e quali fossero i motivi dei continui rinvii che avevano determinato una fortissima preoccupazione nelle realtà industriali segnalate, sia per i posti di lavoro, sia per la sicurezza degli impianti e quindi per la sicurezza degli operai e della stessa popolazione. Con questo mio intervento i senatori firmatari di queste interrogazioni, tra cui io stesso, sollecitano ulteriormente il Ministro dello sviluppo economico ad intervenire e a riferire in Aula.